***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*** «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti, concernenti il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

sull'esito dei lavori della 5a Commissione in relazione ai due maxiemendamenti presentati dal relatore.

Signor Presidente, come prassi, la Commissione bilancio si è oggi riunita e ha attentamente preso in esame

5a Commissione ha preso in attentissimo esame gli aspetti di copertura; purtuttavia, dai colleghi dell'opposizione è stata ampiamente preannunciata una questione di inammissibilità relativa all'intero emendamento 2.0.3000.

si può definire Banca del Sud. Su tale questione i colleghi dell'opposizione non hanno preso in esame il merito (questo

affermando che nella fascicolazione ci sono evidenti errori nella copertura dell'emendamento, perché è stata posta una questione pregiudiziale. Si ritiene, cioè, da parte dei colleghi dell'opposizione, che la materia è inammissibile in Aula, perché il tema non è stato in alcun modo trattato nel corso dell'esame in Commissione bilancio. PRESIDENTE. Sono stati presentati subemendamenti all'emendamento

una questione di pregiudizialità. Il Regolamento, nonché una prassi invalsa continuamente negli ultimi anni, porta, a loro dire, all'inammissibilità di questo testo. Posso naturalmente assicurare lei, signor Presidente, che di questa materia non si era trattato nel corso dell'esame in Commissione. Con riferimento invece all'emendamento 2.3000,

Il Governo, però, su questo punto specifico ha presentato una Relazione tecnica e si è riservato nel prosieguo di fornire i dati analitici richiesti dall'opposizione. Nel suo complesso, sotto i profili di copertura, salvo questa eccezione, l'emendamento è risultato, secondo la Commissione, coperto e di questo si

il criterio univoco al quale si è ritenuto di rifarsi per valutare questo emendamento non è stato quello dell'esatta identificazione di un emendamento elaborato e discusso in Commissione, ma del tema o della materia trattata in sede di Commissione.

Nel passato ormai piuttosto lontano, signor Presidente, qualità e trasparenza della sessione e della decisione di bilancio erano gravemente compromesse dalla possibilità riconosciuta al Governo e al relatore di maggioranza di presentare all'ultimo minuto direttamente in Aula, senza passare attraverso la discussione della Commissione bilancio, proposte emendative che affrontavano questioni del tutto diverse da quelle affrontate dagli emendamenti, magari anche migliaia, esaminati in Commissione. determinava così un grave disordine nella decisione di bilancio, poiché era possibile che argomenti non affrontati e non esaminati adeguatamente entrassero a far parte del del disegno di legge approvato dall'Aula, (del bilancio o della finanziaria o del collegato alla finanziaria) ma soprattutto si determinava una evidente violazione del diritto dei singoli parlamentari dei singoli parlamentari e dei Gruppi parlamentari nel loro complesso rispetto alle prerogative riconosciute al relatore di maggioranza e al Governo. Un parlamentare, se presenta in Aula un emendamento che non ha già presentato in Commissione, lo vede ovviamente dichiarare inammissibile, mentre questa decisione mentre questa decisione non riguardava allora il Governo e il relatore di maggioranza. Durante la legislatura che vedeva presiedere il Senato al collega Pera, sulla base di un dibattito che svolgemmo in Commissione bilancio proprio su questo punto, si addivenne ad una innovazione a mio giudizio molto rilevante. In buona sostanza,

nella legge di contabilità che il Senato, con voto unanime, ha approvato qualche mese fa e che la Camera ha appena finito di esaminare, rinviandoci il testo con modifiche, per un esame che credo comincerà molto presto nella nostra Aula. Si è ribadito, cioè, che ovviamente il relatore ed il Governo possono, anzi, vorrei aggiungere, debbono, su argomenti affrontati in Commissione da emendamenti appositamente preparati, avere il diritto e, per certi aspetti addirittura anche il dovere, di di rielaborare i testi tenendo conto della discussione, ma sempre affrontando questioni o argomenti oggetto di emendamenti presentati in Commissione.

Qualche giorno fa, Presidente, presiedeva il vice presidente Chiti, mi sono rivolto alla Presidenza del Senato al fine di ricordare che, nell'imminenza della presentazione dell'emendamento del relatore, c'era bisogno di ricordare al relatore stesso e al Governo la presenza di questa nostra prassi consolidata, in maniera tale che nel decidere sul contenuto dei suoi emendamenti il relatore potesse aver chiaro qual era il sistema di regole e la prassi consolidata che volevamo seguire e che abbiamo sempre seguito a prescindere dalla maggioranza *pro tempore* del Senato nelle

Noi abbiamo potuto appurare per parere unanime che nessun emendamento, né direttamente né indirettamente presentato in Commissione, affrontava questo problema. Ciò, voglio dirle signor Presidente, non è stato oggetto di controversia, ma è stato riconosciuto pacificamente che nessun emendamento discusso in Commissione aveva affrontato questo tema. Alla luce di questa constatata realtà, giudicata tale da tutti, maggioranza e minoranza, le chiedo, signor Presidente, di dichiarare inammissibile l'emendamento 2.0.3000. emendamento peraltro dovrebbe essere dichiarato inammissibile, a mio giudizio, anche per ragioni di copertura che riassumo brevemente; non le voglio far perdere tempo, ma è importante che si sappia.

ma l'emendamento che all'Aula è stato presentato contiene quelle coperture ed è stato oggetto di subemendamenti da parte di senatori che hanno esaminato l'emendamento che contiene quelle coperture. Naturalmente, anche in Commissione abbiamo dovuto constatare che l'emendamento formalmente contiene quelle coperture, ma l'emendamento, che certamente reca oneri, non è corredato di relazione tecnica in particolare, signor Presidente, su due punti di assoluto rilievo. Il comma 18 dell'emendamento in questione (se lei lo guarda constaterà facilmente che le sto dicendo ciò che è) dispone degli degli sconti fiscali significativi per i percettori di interessi attivi sulle obbligazioni emesse dalla cosiddetta Banca del Sud. Questi sconti fiscali determinano una riduzione di gettito che non è stata in alcun modo quantificata e ancora meno coperta, anche se le ultracoperture previste nel testo dell'emendamento, per gli errori di fascicolazione (per usare l'espressione del presidente Azzollini, di cui ho parlato in precedenza), sembravano recare coperture capaci di corrispondere anche a queste esigenze. Se però quelle coperture vengono espunte dal testo, naturalmente il problema di copertura dell'emendamento esiste e determina, a mio giudizio, una sua inammissibilità. prevede patentemente l'assistenza di garanzie dello Stato sui titoli emessi, senza che sia stata fornita una Relazione tecnica che quantifichi le risorse necessarie per fornire queste garanzie. È inutile che le ricordi, signor Presidente, che negli Stati Uniti d'America due grandi organizzazioni finanziarie fondate esattamente sulla presenza di una garanzia di ultima istanza hanno determinato per il bilancio degli Stati Uniti d'America un buco pari a circa 7.000 miliardi di

il comma 18-*duovicies* e il comma 18-*sexiesvicies* affrontano temi che non erano in alcun modo né affrontati né sfiorati in Commissione. Questo, a nostro avviso, determina l'esigenza di una dichiarazione di inammissibilità di questi due commi. Sottolineo, infine, signor Presidente, che l'emendamento 2.3000 presenta un enorme problema di copertura sul punto che riguarda i 100 milioni relativi alla sicurezza, cioè esattamente il comma

MORANDO *(PD)*. Dell'emendamento 2.3000, di quello che io considero nel suo complesso assolutamente ammissibile. Per quel che riguarda i problemi di copertura, signori colleghi e signor Presidente in particolare, faccio presente la seguente situazione: questo testo utilizza 100 dei 200 milioni disposti come effetto di risparmi recati dalle norme contenute nell'articolo 61 della legge n. 133 del 2008,

Al comma 17, signor Presidente, si stabilisce che le somme provenienti da questa riduzione di spesa vanno a costituire un fondo di 200 milioni di euro;

signor Presidente, risulta scoperta, perché il Governo non ha fornito una relazione tecnica che dimostri che si sono realizzati risparmi che hanno dato luogo al fondo di 200 milioni di cui si sta parlando. Certo, il fatto che il Governo, che ha questi soldi per la sicurezza, ne tolga la metà per finanziare un'altra norma sulla sicurezza fa pensare che in realtà i risparmi non ci siano stati. In ogni caso, questi dovrebbero essere documentati, a pena di inammissibilità dell'emendamento, con una relazione tecnica adeguata. *(Applausi dai Gruppi PD e

degli emendamenti in sessione di bilancio. La circolare del Presidente del Senato del 3 ottobre 2003 aggiunge ulteriori elementi di chiarezza al riguardo. In ultimo, ma non da ultimo, voglio ricordare ai colleghi dell'Aula che i lavori della Commissione bilancio sono stati improntati, con molta serietà e senso di responsabilità, secondo criteri di ammissibilità degli emendamenti che ci sono stati indicati dal presidente Azzollini. Tra questi, primeggiano i criteri di non ammissibilità di emendamenti che abbiano carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. è proprio la fattispecie dell'istituzione complessa della Banca del Sud. Signor Presidente, faccio un appello alla sua sensibilità istituzionale. Se i componenti della Commissione bilancio si sono attenuti rigorosamente

prerogative, delle facoltà di tutti i parlamentari, di fronte alle funzioni e alle competenze dell'Aula del Senato. Signor Presidente, spiace constatare che proprio il PD, che ha come Capogruppo

come tante persone ed imprese del Sud che aspettavano questo momento, di come proprio il PD ne impedisca non soltanto l'approfondimento, il dibattito e l'eventuale miglioramento in quest'Aula,

Prendiamo atto che ancora una volta il Partito Democratico dice alle piccole e medie imprese del Sud di continuare ad aspettare. Il Governo Berlusconi vuole lo sviluppo del Sud e lo dimostra; vuole fatti, mentre c'è qualcun altro che fa soltanto chiacchiere. Assistiamo in questi ultimi giorni soprattutto ad una politica di fogli lanciati contro il muro. Ieri no, oggi ancora un altro no. Penso che sia un ostruzionismo miope

*(PdL)*. So che certi argomenti probabilmente non sono ben accetti, ma non è con l'ostruzionismo e con i cavilli regolamentari, senatore Morando, che diamo risposte al Meridione. proprio con questo ostruzionismo miope che bisogna far pesare allo sviluppo del Sud e alla pelle delle persone che vi abitano la necessità di una politica di crescita. Tutti invocano a parole una soluzione, una risposta seria e concreta e una politica incisiva di crescita. Invece voi vi attaccate a cavilli regolamentari per non assumervi le vostre responsabilità politiche, e pur di non riconoscere i meriti al presidente e al Governo Berlusconi voi mandereste a picco non soltanto il Meridione ma l'Italia intera.

sulla proposta del Governo, trincerata dietro l'emendamento del relatore presentato all'Assemblea, non perché sia inammissibile ma perché nel merito, politicamente, non serve al Mezzogiorno

dell'emendamento, come lei avrà notato, perché credo che sarebbe più interessante, anche per i Gruppi parlamentari di opposizione, affrontare questo argomento, disponendo di accorgerci poi che si tratta dell'ennesima bufala che rinvia ad una decisione dell'Unione europea su come, quando e in che termini affrontare il tema del credito nel Mezzogiorno, cosa diversa dalla Banca del Sud e da tutto questo

è caduta in particolare sull'osservazione del senatore Morando che, in buona parte, coincide con le sue osservazioni sulle presunte inammissibilità. Lei ha sollevato l'inammissibilità presunta del comma 18-*duovicies*, mentre il senatore Morando ha aggiunto qualche perplessità anche sul comma 18-*sexiesvicies*, sul tema del fondo per giustizia e sicurezza proveniente dai beni confiscati.

Non era questa la domanda, stiamo parlando di inammissibilità,

con un'interpretazione anche estensiva, a materie trattate in Commissione bilancio. Il Regolamento parla di proposte emendative, ma, volendo, possiamo interpretarlo anche con riferimento a materie trattate analoghe ai nuovi emendamenti.

non è stato nemmeno sfiorato il tema, né attraverso emendamenti né attraverso ordini del giorno, per cui va dichiarato inammissibile.

la messa a reddito di tutti i beni ed immobili confiscati alla criminalità organizzata che servono a finanziare un Fondo unico a favore

Tecnicamente il Regolamento mi impone, per quel rispetto delle regole alle quali io quotidianamente cerco di ispirarmi, la dichiarazione di inammissibilità e devo farla a malincuore, ma con quel rigore che mi sono imposto: l'argomento non è stato trattato in Commissione e l'emendamento va quindi dichiarato inammissibile. Questo argomento

a migliorare ed amplificare quel dibattito tra le parti, tra maggioranza e opposizione, al quale sempre mi richiamo. Mi spiace che in questa occasione né la Commissione, in sede di esame del maxiemendamento, né l'Assemblea abbiano la possibilità di potersi confrontare. sono mai stato - credo che mi si debba dare atto di ciò - fiscalissimo nella concessione dei tempi e sarei stato pronto a dare alla Commissione ulteriori tempi per discutere questo subemendamento, che è formalmente inammissibile, se vi fosse stata la volontà di tutte le parti di in deroga, ammissibile, ma soltanto dietro una condivisione. Questa condivisione non c'è. Prendo, quindi, atto dell'obiezione procedurale del senatore Morando, la ritengo fondata nel merito, per cui dichiaro inammissibile l'emendamento 2.0.3000 sulla Banca del Sud. Di

Apparentemente si assegnano 100 milioni di euro al personale della Polizia di Stato, ma, con un comma successivo, si sottraggono 100 milioni di euro al fondo istituito e destinato alla tutela della sicurezza pubblica, inclusa l'assunzione di personale. cioè, di una presa in giro: sono 100 milioni di euro che si spostano all'interno del dipartimento e che riguardano sempre il personale.

100 in più da una parte, 100 in meno dall'altra, il risultato è zero. Se vogliamo dare 100 milioni al personale dobbiamo darne 200, perché poi ne togliamo 100 dall'altra parte. Ecco la ragione del nostro subemendamento, non si può girare pagina e trovare la negazione di quello che si è affermato nella pagina precedente. Sarebbe stato forse formalmente più corretto

abbastanza risibile, se non fosse drammatico, quello che state facendo. Il mio emendamento cerca pertanto di porre rimedio a questa farsa.

in favore della tecnologie avanzate, dell'efficienza energetica e della tutela ambientale in riferimento ad alcune Regioni. Sono infatti comprese tutte le Regioni del Mezzogiorno:

nell'istituzione della Banca del Sud il relatore, e quindi penso anche il Governo in quanto ha espresso parere conforme, ha considerato le Regioni del Mezzogiorno comprensive anche di Abruzzo e Molise. Invece, in questo emendamento in cui si prevedono contributi per l'incentivazione della ricerca, della tutela ambientale e delle tecnologie avanzate, per una discrepanza e una discordanza, mancano le due Regioni Abruzzo e Molise. che si tratti semplicemente di una svista e pertanto chiediamo al relatore di poter esprimere un parere favorevole nei confronti di tali emendamenti correttivi, anche perché non pensiamo che i parlamentari di quelle Regioni siano meno attenti e sensibili di quanto lo siano i rappresentanti di tutte le altre Regioni del Sud. 2.3000 (testo 3)/11. Il CNR dà un contributo prezioso alla ricerca e allo sviluppo competitivo del nostro Paese. Per questo motivo ci pare quantomeno strano che si voglia affidare al CNR il compito di coordinare progetti di promozione industriale per la cui attività esistono altre strutture che hanno realizzato sul campo una significativa esperienza. è necessario consolidare la rete dei presidi CNR nel Mezzogiorno. Per questo motivo noi proponiamo, considerato che i temi di cui si parla sono esattamente quelli di cui si è occupato il programma strategico «Industria 2015», per il quale esistono proposte d'intervento industriale nel Mezzogiorno d'Italia non finanziate per carenze di risorse finanziarie, di collocare di collocare su quelle azioni le necessarie risorse finanziarie perché gli investimenti possano essere sostenuti con gli strumenti del regime di aiuti vigente nel nostro Paese. Proponiamo, al tempo stesso, di potenziare la rete del CNR mettendo a disposizione dello sviluppo industriale e dei progetti di insediamento industriale nelle Regioni del Mezzogiorno la propria attività di ricerca la propria attività di ricerca e di verifica anche precompetitiva dei risultati della ricerca conseguiti nel corso di questi anni.

di strutture che svolgono una funzione di straordinaria efficacia e importanza nella lotta al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Sappiamo tutti quanto questo sia un punto di sofferenza, un nervo scoperto circa l'andamento delle entrate e come sarebbe importante aggiungere una capacità di operatività migliore, soprattutto andando a dare una risposta a un paradosso. Ci sono, infatti, graduatorie che sono tuttora valide di persone che hanno maturato il diritto a essere assunte, ma che senza quelle risorse finanziarie rischiano di vedersi negati

caso viene il sospetto, signor Presidente e signor vice ministro Vegas, di un gioco delle tre carte che il Governo è abilissimo a fare.

dell'imprenditorialità e dell'occupazione tra i giovani, ma poi si attingono le risorse abrogando un fondo che era disposto proprio per sostenere e finanziare l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, era riconducibile all'accordo fatto

Vorrei ricordare a tutti colleghi, che prego di fare un attimo di attenzione, che sono trascorsi ormai cinque mesi dalla data del disastro ferroviario che ha colpito Viareggio. Puntualmente, ogni 29 del mese, tutta la città si mobilita per ricordare con forza quanto è accaduto e quanto è dovuto moralmente e materialmente alla nostra città e ai nostri concittadini colpiti dal tragico evento. Dopo la nomina del commissario straordinario, dopo attente e ponderate valutazioni, è emersa chiaramente l'assoluta insufficienza dei fondi stanziati dal Governo non solo per i danni materiali ma anche e soprattutto per l'indennizzo e il sostegno di complesse situazioni familiari. Ricordo ai colleghi che interi nuclei familiari sono stati distrutti e che, a seguito di questo disastro, molte persone, per lunghissimo tempo, non potranno più badare ai propri congiunti. Ad oggi, i vari ordini del giorno approvati dalle Assemblee non hanno trovato alcun seguito da parte del Governo. Le proposte di legge non sono state ancora messe in discussione. Le indagini si annunciano ancora lunghe e complesse mentre le vittime hanno ricevuto solo minime forme di indennizzo, peraltro finanziate da libere elargizioni e dallo stanziamento della Regione Toscana. Sulla stampa compare poi la possibile intenzione da parte delle Ferrovie e della GATX di anticipare i risarcimenti, ma niente di concreto. Su tutto aleggia ancora un'aria di incertezza che concorre a demoralizzare ancora di più le persone colpite da una calamità giustamente definita innaturale perché causata dall'incuria e dalla mancanza di sicurezza. Nello stesso tempo giova ricordare che l'INPS di Lucca, giustamente, chiede e promette azioni di recupero nei confronti di aziende che peraltro sono state chiuse, danneggiate o completamente distrutte.

in attesa dell'accertamento delle responsabilità, siano l'ente gestore delle Ferrovie e le società coinvolte ad anticipare le risorse dovute.

sottolineava l'importanza e la nobiltà del provvedimento. Presidente, sono "costretto" a dirle che c'è un inganno, perché la soluzione proposta è quella della vendita dei beni confiscati alla mafia. *(Brusìo. In tutti questi anni, ci siamo divisi sulla lotta alla mafia; su un punto, però, pensavo che potessimo continuare a mantenere un filo di unità, ed era l'esclusione della vendita dei beni confiscati. Lo abbiamo detto in tante occasioni, anche solenni e istituzionali. In Commissione antimafia ci sono numerosi documenti

e un po' improvvido, si apre una maglia su un sistema che invece avrebbe bisogno di ben altri interventi, come ad esempio la costituzione moderna e avanzata di un'agenzia specializzata, per sottrarre all'Agenzia del demanio una funzione che - è stato dimostrato - non è in grado di espletare al meglio. Ecco perché, Presidente, ho voluto prendere la parola, perché se sui beni confiscati apriamo la maglia della vendita, come lei ben sa, ciò significa sottoporci ad una pressione e ad un'incursione da parte delle mafie che sarebbe bene evitare.

che emerge dal comma 18-*sexiesvicies*. Illustro in particolare il subemendamento 2.3000 (testo 3)/38, che fa riferimento sostanzialmente al Fondo unico giustizia.

tutte le somme di denaro sequestrate e i proventi derivati dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o misure di prevenzione; una parte doveva essere destinata alla sicurezza pubblica e un'altra al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. Questa idea di autofinanziare la giustizia è sicuramente seria e condivisibile, però quello che sta succedendo è esattamente il contrario. In pratica, il Governo, attraverso l'emendamento del relatore, vorrebbe farci credere che con questa legge finanziaria il Fondo unico giustizia verrebbe implementato. Questo non è assolutamente vero, è una presa in giro, perché con questo emendamento voi svuotate, anche formalmente, il Fondo unico per la giustizia, perché disponete che le eventuali risorse, delle quali abbiamo chiesto contezza ripetutamente da dieci mesi al Ministro della giustizia in Commissione, non siano destinate direttamente al Ministero della giustizia e a quello dell'interno, ma finiscano nel grande calderone del ministro Tremonti, con buona pace del Fondo unico giustizia, riservato appunto a sicurezza e giustizia.

un tempo che almeno arrivi fino al 31 dicembre, un anno. Qui siamo alla farsa: prima ci è arrivata una proposta senza alcuna copertura di spesa e senza un'indicazione del costo dell'operazione; poi questa è stata rivista e si è

per coprire questa spesa si usi sempre la stessa coperta. Si vanno a togliere risorse sul bioetanolo e sul biodiesel: è grave per l'ambiente, ma oltretutto sono risorse collegate ai processi di riconversione degli ex zuccherifici.

abbiate il coraggio di comunicare ai consorzi di garanzia, che proprio sulla scorta delle vostre promesse hanno anticipato la quota pubblica per la fine del 2008-2009, che a dicembre dovranno dire ai produttori che non era vero niente e che dovranno farsi carico loro per il futuro degli altissimi costi legati ai rischi climatici, costi che per le imprese diventano enormi. Abbiate finalmente il coraggio di dire che per voi l'agricoltura è l'ultimo dei vostri pensieri, avendo però nel contempo la decenza di non dire che questi maxiemendamenti, questi provvedimenti che stanno rimbalzando tra le due Camere,

e hanno una scadenza. Chiedo semplicemente di chiarire una volta per tutte che i lavoratori frontalieri non sono assimilabili ai delinquenti e agli evasori fiscali, ma si tratta semplicemente del loro stipendio. caso, cari amici della Lega, non sto parlando di cittadini elettori che risiedono nel mio collegio, ma di cittadini che risiedono nel vostro collegio. Lasciate passare questa disposizione e li incoraggerete a diventare rapidamente dei vostri ex elettori: di questo non posso che ringraziarvi.

Basta una lettura del testo per comprendere che i 200 milioni che erano contenuti in quel comma e che sono stati versati in bilancio possono essere utilizzati. Altrimenti non si sarebbero potuti versare in bilancio. È l'eventuale esubero di questa cifra che va in economia su cui si può eventualmente discutere. 200 milioni sono assicurati al bilancio, altrimenti non si sarebbero potuti utilizzare e la relazione tecnica fornita dalla Ragioneria sarebbe stata contraria.

una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale (...)». La norma del comma in esame, il 18-*sexdecies*, in realtà consente una cosa leggermente diversa, che è l'utilizzo

«Difesa Servizi Spa». Ieri quest'Aula ha confermato il proprio voto a favore di questa Agenzia che privatizza di fatto l'Esercito italiano e le Forze armate. Il nostro emendamento tendeva a sottrarre almeno la gestione degli immobili, cosa che invece mi pare voglia essere concessa ulteriormente dal Governo in carica. riguarda la concessione di altri 100 milioni di euro alle forze di polizia e al comparto difesa e sicurezza. La puntualizzazione che ha fatto il Vice Ministro non ci convince. Di fatto, anziché dare 100 milioni ...

della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

Presidente, vorrei segnalare la gravità dell'intervento che si attua con questa normativa. Viene azzerato il settore dell'incentivazione ai carburanti ecologici. Tutti i Governi intervengono sull'economia verde e questo Governo provvede ad azzerare l'intervento sul bioetanolo (si passa da un'incentivazione di 73 miliardi a 4 milioni di lire) e ad azzerare l'intervento per il biodiesel da 250.000 tonnellate agevolate a 18.000, aumentando dell'80 per cento l'accisa. Si tratta di aziende che hanno investito. È incredibile che il Governo possa fare questo. Mi auguro che nel passaggio alla Camera si trovi una diversa copertura e si ristabilisca l'incentivazione in un settore strategico com'è quello dei carburanti ecologici.

che le elargisca pure, ma senza farle passare per un beneficio al Sud dell'Italia!

esiste il programma "Industria 2015", su cui centinaia di imprese hanno presentato progetti integrati tra istituti di ricerca pubblici e privati e aziende, esattamente nelle materie che sono previste in questo provvedimento. Come è possibile finanziare un ente pubblico per futuri progetti di ricerca, quando sono pronti ed eseguiti, sulla base di una promessa dello Stato, progetti che si tradurrebbero immediatamente in attività? Dunque, finanziamo i progetti previsti dal programma "Industria 2015" ed eventualmente sosteniamo anche il CNR. Ma prima finanziamo quelli.

Se non si interviene immediatamente con un defibrillatore, la mortalità è altissima, soltanto due persone su cento si salvano. Se si interviene con un defibrillatore,

mettendo i defibrillatori in tutti i luoghi pubblici, a cominciare da quelli dove si svolge attività sportiva. È un calcolo che abbiamo fatto insieme, in Commissione sanità, nella passata legislatura, perché questa legge venne presentata da Forza Italia e il relatore fu il presidente Tomassini. Credo che sia difficile avere un rapporto costo‑beneficio migliore di questo: aumentare lo stanziamento di 2 milioni e arrivare a poter salvare...

Prego, senatore che dovrebbe dare avvio ad un programma straordinario per la difesa del suolo. Oggi Governo e maggioranza esprimono parere contrario su questi subemendamenti che vanno nella stessa direzione. Tutto questo avviene dopo che gli ultimi tre o quattro mesi hanno confermato l'altissimo tributo di vite umane che il nostro Paese paga al dissesto idrogeologico del territorio. La domanda che rivolgo al Governo e alla maggioranza è quanti altri morti dovremo aspettare, prima che il Governo Berlusconi e la maggioranza che lo sostiene si decidano ad impegnarsi su questo fronte, che è decisivo per il benessere di tutti i cittadini.

cittadini. L'impossibilità di trovare in una manovra finanziaria come questa le risorse da funzionalizzare in via esclusiva a questo tipo di intervento ci sembra obiettivamente di pessimo

appello a lei, signor Presidente, e ai colleghi della maggioranza perché ritengo che su questo argomento sarebbe opportuno che il Senato desse un segnale di pronto intervento diretto alla città e alle vittime, così come pronto è stato l'intervento delle istituzioni in occasione della tragedia. Con

Sono stato tra coloro i quali hanno plaudito alla visita del Presidente del Consiglio il giorno immediatamente successivo alla disgrazia immane che ha colpito questa città toscana. Impegni precisi sono stati assunti e mi auguro che questo Parlamento nella giornata odierna, con l'approvazione di questo emendamento, voglia dare seguito a quegli impegni presi dal Governo e, quindi, dalle istituzioni italiane.

più volte sollecitato al Governo nei diversi esponenti che si sono succeduti in Aula e ai relatori, come la rappresentazione più evidente della disattenzione e della più completa assenza di interlocuzione tra il Movimento per le Autonomie, il Governo e la maggioranza. Questo emendamento fa pagare ad un piccolo comparto produttivo di un piccolo comprensorio meridionale l'inefficienza di una burocrazia ministeriale che ha sbagliato a scrivere due ordinanze di protezione civile facendo confusione tra meccanismi contributivi e meccanismi tributari. Adesso, in una fase di crisi, questo errore diventa un gravame pesantissimo per quelle piccole aziende, ma la totale disattenzione ha impedito in quest'Aula che si potesse porre riparo e rimedio a questa vicenda. Ne prendo atto.

ad un interessante dibattito - devo dire *bipartisan* - tra il presidente Baldassarri ed il senatore Rutelli sulla cedolare secca del 20 per cento. Questo emendamento si propone di introdurre la cedolare secca per le locazioni nel Comune dell'Aquila che interessano gli studenti universitari. C'è stato un appello pubblico del rettore dell'università per il fatto che gli studenti stanno emigrando dalla sede universitaria per l'impossibilità di trovare degli alloggi. Con questo emendamento si ottengono due obiettivi: da un lato si stimola la locazione e dall'altro facciamo anche un piccolo laboratorio sperimentale sui saldi di finanza pubblica

Signor Presidente, beni confiscati alla mafia: si apre la maglia delle vendite. Pensate un po', colleghi, che questa vendita viene messa nelle mani del dirigente del competente ufficio del territorio (sottolineo, territorio) dell'Agenzia del demanio. Pensate un po', un dirigente a 3.000 euro al mese che deve, nel territorio, contrastare la possibilità delle mafie di comprarsi un bene del valore di 200 milioni di euro. Pensate che scelta scellerata il Governo oggi ci propone. Ecco perché chiediamo al Governo di ripensarci, di ritirare questa ipotesi, di riorganizzarla in un altro modo e di fare bene la propria attività di tutela e di messa a reddito dei beni confiscati.

si può fare l'assegnazione dei beni confiscati attraverso l'Agenzia del demanio: è una pura follia ed è un modo ipocrita per non fare queste operazioni. Insistere anche in questa finanziaria su questi aspetti, quindi, è demenziale ed irresponsabile.

di esecuzione per la revoca della confisca. Pensare che l'Agenzia del demanio territoriale possa gestire un 30 per cento di questi patrimoni con una massa di occupanti abusivi è fuor di logica. Significa non dare nulla alla giustizia.

Presidente, l'emendamento in esame vuole contribuire a migliorare l'utilizzo di queste risorse derivanti dalle confische. Non si può limitarne l'uso alla copertura degli eventuali buchi di bilancio determinati da esigenze di cassa definite dal Ministro dell'economia con i tagli lineari, resi anche ai Ministeri impegnati nelle politiche di ordine pubblico, di sicurezza e contrasto alla criminalità. Le confische gravano su territori che pagano il prezzo dell'aggressione mafiosa. Desidero che questo emendamento sia valutato con apertura perché pretende soltanto che la parte prevalente di queste risorse sia utilizzata per rafforzare operativamente tutte le strutture giudiziarie e di polizia che operano nei territori in cui è avvenuta confisca. risorse rimangono nell'ambito di quell'amministrazione ma con una finalizzazione precisa nei territori in cui la confisca è avvenuta. Chiediamo Signor Presidente, chiedo al collega Pistorio se è d'accordo che io apponga la mia firma. Voglio sottolineare che il ministro Alfano, circa un mese fa, proprio su questo tema, intervenendo ad un convegno sui beni confiscati alla mafia, disse che era necessario intervenire normativamente per dare un indirizzo affinché i beni confiscati e i proventi fossero reimpiegati nelle stesse Regioni dove sono stati confiscati. Per questa ragione, credo sarebbe opportuno accogliere la proposta del collega Pistorio.

solo sui tartufi. L'agricoltura italiana ha bisogno di soldi veri e non di bufale metropolitane, per le quali evidentemente per questa maggioranza dovremmo richiedere il marchio DOC.

accise è una battaglia storica; non piacerà, ma è una nostra battaglia. Vorremmo che una quota limitata delle accise sui prodotti che vengono raffinati nel nostro territorio, e che inquinano pesantemente, fosse utilizzata per finanziare un piano di riassetto idrogeologico ad un'emergenza denunciata a tutti i livelli. Vorremmo provvedere con una parte di risorse che vengono a realizzarsi a seguito dell'utilizzo sul territorio di quelle attività fortemente inquinanti.

Il vice ministro Vegas, nell'illustrare il suo parere, ha riferito che dal punto di vista del Governo non sarebbe necessaria una norma di tal genere per eliminare un'anomalia che si sta verificando. In realtà, le cose non stanno così, almeno allo stato, nel senso che, come ha detto e scritto il collega Micheloni, i lavoratori italiani transfrontalieri sono stati raggiunti da un invito-diffida dell'Agenzia delle entrate per assoggettare i redditi da lavoro e da pensione, sui quali assolvono le imposte, allo scudo fiscale. È uno scandalo, signor Presidente. Allora, o il Governo consente di introdurre questa norma interpretativa, che è assolutamente doverosa, o, in caso contrario, accolga un ordine del giorno - in questo caso lo chiediamo noi - che sia però effettivamente impegnativo, non nel senso di emanare, chissa quando, una norma chiarificatrice, ma nel senso di impegnare il Governo ad invitare, con atto cogente, l'Agenzia delle entrate a ritirare la circolare,

sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che l'ho detto. Adesso introduciamo la categoria dell'ordine del giorno impegnativo, che va bene per la circostanza *de qua*, ma - ripeto - io sono assolutamente d'accordo. Il problema si può risolvere con un ordine del giorno, non è necessaria una norma legislativa. Quindi, se l'emendamento

siccome siamo in prossimità del ritocco del canone RAI, si evoca il fatto che il medesimo canone RAI può essere lievemente innalzato anche per far fronte alle necessità di investimento delle reti locali sul digitale. Pregheremmo, quindi, di

sulla legge finanziaria, non ho fatto mancare il tono della mia voce come contributo appassionato a questo lavoro parlamentare del quale si coglie ogni giorno di più l'assoluta inutilità. Francamente, partecipare con la massima convinzione, per fede nella cultura parlamentare, a questo impegno che dovrebbe essere tra i più rilevanti della vita politica e dover assistere,

Accanto a ciò, si deve prendere atto della totale disattenzione che la maggioranza di Governo

i parlamentari e l'Esecutivo. Ebbene, per quanto ci riguarda, abbiamo preso atto che questo non si è realizzato in alcun modo e che nessuna nostra proposta, da quelle

Abbiamo anche preso atto di un umore montante di insofferenza ulteriore per le Regioni del Mezzogiorno, che probabilmente abbiamo il torto di rappresentare male, ma questo è il nostro dovere e lo faremo con ancora più convinzione. convinzione. Io denuncio ‑ lo dico agli amici Capigruppo del PdL, Gasparri e Quagliariello - che vi è una difficoltà politica molto seria nel rapporto di maggioranzatra il Movimento per le Autonomie e il

critica, che rendiamo esplicita in questa occasione non votando la legge finanziaria. Il voto del Movimento per le Autonomie sarà di astensione, che al Senato vale come un voto contrario. È un atto esteticamente meno aspro, ma nella sostanza è una presa di distanza da questo provvedimento, non solo per quello che ha determinato in termini di relazioni politiche ma anche per il contenuto totalmente disattento al tema del Mezzogiorno, che doveva essere affrontato enfaticamente con l'ipotesi, tutta da verificare, della Banca del Sud; un emendamento che, per ragioni procedurali, è venuto meno senza

dello sviluppo del Sud, quindi anche in ragione del venir meno dell'emendamento del relatore che doveva consentire quantomeno il dibattito su quello strumento straordinario che era la Banca del Sud, annunciamo il voto di astensione del Movimento per le Autonomie sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

poiché la gravità, l'enormità e l'inutilità di ciò che la maggioranza si appresta a votare sono così grandi, per un atto di riguardo nei confronti di chi ci ascolta e del Parlamento, credo sia giusto dare una motivazione articolata al nostro voto contrario ad un provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, sarà inutile rispetto all'andamento economico e alla situazione sociale del nostro Paese. Non più tardi di due mesi fa, signor Presidente, abbiamo rilevato come il Documento di programmazione economico‑finanziaria registrasse un pesante crollo dei consumi e della domanda nel nostro Paese, con un pericoloso ridimensionamento dei redditi reali e del potere d'acquisto delle nostre famiglie. Tutte conseguenze, sì, dell'impatto enorme della crisi economica, ma anche inevitabile frutto del pesante effetto leva che la crisi ha generato a causa della carenza nel nostro Paese di un sistema di mercato del lavoro, economico e istituzionale adeguato, o almeno lontano dallo scadente*status* in cui riversa, se messo a confronto con i principali Paesi europei. Sempre in occasione di quella discussione, abbiamo preso atto della circostanza che alla fine del 2008 si rilevava una diminuzione del 13,5 per cento rispetto al 2007 della ricchezza finanziaria netta in possesso delle famiglie italiane. In aggravio a tale condizione di indubbio svantaggio per i cittadini, abbiamo anche evidenziato come, soprattutto negli ultimi mesi, la qualità del credito ad imprese e famiglie si sia deteriorata, comportando un aumento del rapporto tra sofferenze e credito concesso. In parole povere, aumento della povertà degli individui e delle imprese, costrette a chiudere. Particolarmente deprimenti sono poi le condizioni del mercato del lavoro, che ha visto produrre, parole recenti del governatore Draghi, solo quest'anno un aumento di 650.000 disoccupati sull'intero panorama nazionale. Questa è la fotografia sbiadita del Paese in cui viviamo. Questi i concetti che dovremmo tenere tutti bene impressi, soprattutto ora che quest'Assemblea si trova ad approvare l'ennesimo provvedimento economico, questa volta quello madre, la finanziaria, senza aver benché minimamente offerto segno tangibile di una percezione, o almeno qualcosa che vagamente le somigli, della realtà del nostro Paese e delle condizioni disastrose in cui si trovano gli italiani. È vero, i primi segnali di ripresa sottolineati dall'aumento del prodotto interno lordo dell'ultimo trimestre ci fanno ben sperare, ma il rischio forte è che si tratti solo di segnali non destinati ad avere una forte continuità. Il nostro è un Il nostro è un Paese fermo, o meglio sta cercando lentamente di rialzarsi e riprendere a camminare grazie alla passione della gente ed alla volontà di non mollare, ma non può che farlo con fatica e con il freno a mano tirato, in nome di un passato ma soprattutto di un presente politico profondamente miope di fronte alle reali necessità che andrebbero affrontate per risollevarne le sorti. Il relatore sottolineava non a torto come, a suo dire, la nostra spada di Damocle fosse il debito pubblico. Indubbiamente questo è vero, ma è altrettanto vero che è arrivato il tempo di scelte convinte, serie e difficili. È arrivato il momento di comprendere che se non si offrono risposte concrete a famiglie, lavoratori ed imprese, il nostro Paese è destinato a diventare ancor più di quanto non sia già la Cenerentola d'Europa o, se preferite, il carrozzone d'Europa. Eppure l'occasione, colleghi, era propizia. Il Governo, favorito anche da una buona dose di mancanza di coraggio e volontà da parte della maggioranza rappresentata in quest'Assemblea,

sul quoziente familiare; sull'aumento delle detrazioni per oneri di famiglia; sulla trasformazione delle detrazioni per oneri di famiglia in deduzioni; sull'aumento degli assegni familiari, sul contributo per i genitori che intendano diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura del figlio nato; sull'aumento del 10 per cento dell'importo massimo di detrazione degli interessi passivi sui mutui per ciascun figlio a carico; sulla detraibilità delle spese per l'acqua, per la luce e per il gas per i contribuenti con tre o più figli a carico; sull'aumento della detrazione delle spese mediche per i contribuenti con figli a carico; sul contributo a favore dei figli minori frequentanti scuole paritarie a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche; sulla detraibilità delle spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria, comprese le spese per l'acquisto dei testi scolastici; sui contributi dei figli frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado; sulla deducibilità delle spese fatturate di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relativa agli immobili, il cosiddetto contrasto di interessi. nato; sull'aumento del 10 per cento dell'importo massimo di detrazione degli interessi passivi sui mutui per ciascun figlio a carico;

della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di scuole materne paritarie, primaria e secondaria di primo e secondo grado per i figli. Sull'incremento di 30 milioni di euro per il capitolo Fondo scorta per la Polizia di Stato e quant'altro, sulla cedolare secca e su tutti gli altri emendamenti. Non c'è un solo intervento, piccolo, medio o grande, a sostegno delle famiglie italiane che la maggioranza ed il Governo abbiano assecondato ed approvato. Non vengano a raccontare chiacchiere: non c'è alcun intervento che riguardi il sostegno alle piccole e alle medie imprese. Si è partiti con il taglio dell'IRAP annunciato dal presidente Berlusconi all'assemblea di Confartigianato; si è passati al taglio dell'IRAP per le piccole e medie imprese; si è passati poi alla deducibilità solo per le imprese che avessero bilanci in perdita; si è arrivati, quindi, al taglio dell'IRES e ieri sera si è giunti alla partita di giro truffaldina sullo sconto del 20 per cento sull'acconto IRPEF di fine anno per i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi e le partite IVA.

di utilizzarla invece coprendo ora il buco relativo al taglio dello sconto sull'acconto IRPEF, recuperandolo con l'extragettito nel 2010. In altri termini, i contribuenti italiani che oggi pensano di avere avuto il taglio delle tasse e che spenderanno i loro soldi a Natale, ripagheranno con gli interessi al fisco quello che non hanno pagato in termini di acconto nel 2009 e lo ripagheranno nel 2010 anche con l'aumento del debito pubblico. Questo è il miracolo italiano che il Governo sta ammannendo a noi e alle nostre famiglie! Inoltre, signor Presidente, credo che non possiamo non fare un'analisi impietosa di una finanziaria che non c'è qui, al Senato. In questo ramo del Parlamento la finanziaria non c'è per due ragioni: innanzi tutto, non vi sono i fondi per le coperture e, quindi, si tratta di una manovra fallace, di un effetto *spot* e di misure che non hanno alcun tipo di rilievo; in secondo luogo, bisogna liberare il Senato da argomenti da trattare perché c'è la "questione madre" che la prossima settimana troverà l'ingresso nelle aule della Commissione giustizia e di cui ci dobbiamo occupare. Il nostro Paese, infatti, non si deve occupare del taglio delle spese inutili, degli incentivi alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori al sostegno di chi si trova in condizioni peggiori; si deve occupare di tagliare alcuni processi! Questo moralmente, ancor prima che politicamente, è assolutamente inaccettabile per ogni cittadino per bene del nostro Paese! *(Applausi dai Gruppi

da alcuni colleghi di maggioranza con grande onestà intellettuale con i loro emendamenti, trovi alla Camera dei deputati quel giusto sostegno che serva a far uscire il nostro Paese dall'immobilismo di un Governo che non si occupa dei problemi reali dei cittadini italiani

Nelle pagine della storia o meglio nei verbali di seduta resteranno scolpite le parole del vice ministro Vegas, che sulle nostre proposte che tentavano di fornire una risposta ai tanti problemi irrisolti del nostro Paese,

Così abbiamo appreso, in una novella riscrittura della Costituzione materiale, che il Senato è l'anticamera della Camera. Un epilogo d'altronde che era già stato annunciato dai titoli di apertura del TG1 di Minzolini di una settimana fa: «Ripresa economica in forte slancio. L'Italia è il sesto paese più ricco del mondo». Seguiva la dichiarazione autocelebrativa e senza contraddittorio del ministro Tremonti, che dichiarava: «Il tempo è stato galantuomo. Non si cambia nulla. Bisogna insistere». È difficile, cari colleghi, insistere sul nulla. Dopo mesi di chiacchiere, *gossip* e sciaguratezze avremmo voluto tornare ad affrontare in modo serio i problemi del nostro Paese e invece ci parlate di un nuovo miracolo italiano. Non abbiamo bisogno di spiegare ai molti italiani che vivono con redditi iniqui, con una pensione indecente o l'incertezza di un lavoro oggi per il domani, che il super indice OCSE è soltanto una statistica, derivata da altre statistiche, che indica una probabilità e che la stessa OCSE invita alla cautela. cautela. Cari colleghi della maggioranza, non avete saputo o voluto fare altro che presentarci una finanziaria in cui l'unico aumento è quello delle promesse, l'unico calo è quello degli aiuti. Una finanziaria in cui tra un emendamento e l'altro ci avete proposto tutto e il contrario di tutto: dalle detrazioni fiscali per i raccoglitori occasionali di tartufo alla riduzione delle accise per il gasolio delle imbarcazioni di pesca a Lampedusa. Oggi abbiamo il dovere di dire agli italiani che una maggioranza di centrodestra confusa e contraddittoria è più in crisi della stessa crisi. Signor Presidente, vi sono almeno 10 buone ragioni per cui non voteremo questa finanziaria. Molte sono le domande a cui abbiamo voluto dare delle soluzioni con i nostri emendamenti e troppe le questioni irrisolte. Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio un posto fisso o un precario? Noi vi abbiamo risposto che è una vergognosa presa in giro parlare di posti fissi in un Paese che al momento non produce neppure posti precari. Noi abbiamo chiesto al Governo di mettere da parte i colpi di teatro e gli effetti annuncio e di affrontare i problemi vissuti da milioni di italiani, tutelando le fasce sociali non coperte, rendendo più uniformi le protezioni, creando un percorso di ingresso al lavoro con regole nuove, per conciliare flessibilità e tutela. Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio pagare l'IRAP o abolirla? Noi diciamo che sarebbe un delitto non fare nulla, rinviando al futuro la riduzione IRAP sul costo del lavoro e sul costo degli interessi, perché le imprese hanno un bisogno urgente di questo aiuto, oggi più di domani, per il semplice fatto che domani molte rischiano di essere ex imprese. Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio continuare a far pesare sui comuni il debito pubblico o continuare soltanto a parlare di federalismo delle autonomie? Riteniamo che il Patto di stabilità, con la misera modifica dello sblocco del 4 per cento, insieme alle minori entrate, rendano la situazione dei Comuni drammatica, con una perdita di entrate di oltre 1 miliardo di euro. Voi della maggioranza vi siete chiesti: meglio i Tremonti Bond, che nessuno ha voluto, o una diversa politica di sostegno alle piccole e medie imprese? Noi diciamo che detassare gli utili reinvestiti quando non se ne fanno o limitarli a poche categorie, ridurre i fondi per la ricerca e innovazione, applicare sull'accesso al credito d'imposta il *click day*, che ha già esaurito al 2008 l'intero stanziamento fino al 2015, non aiuti la competitività e la sopravvivenza delle nostre imprese, siano esse del profondo Sud, siano esse del Nord, della Padania. Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio impegnare risorse come i 3 miliardi per difendere la compagnia aerea di bandiera o tutelare la famiglia che significa, quella sì, salvaguardare la coesione e la tenuta della nostra società civile? Noi diciamo che la politica dei tagli non va fatta pagare alle famiglie italiane. In due anni di Governo di centrodestra le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni sono diminuite di due terzi e tra queste mancano all'appello i 400 milioni per la non autosufficienza i 100 milioni per la prima infanzia e lo stesso Fondo nazionale per le politiche sociali sarà ridotto alla risibile somma di 140 milioni. Avete prodotto, di fatto, una controriforma, facendoci passare dallo Stato sociale allo Stato minimo. vi siete chiesti: è meglio una banca del Sud o continuare semplicemente a parlare del Sud come questione nazionale? Noi riteniamo che non si tratta di fare una nuova banca cui dietro un aggettivo si nasconde un ritorno ai vecchi metodi del passato, o costruzioni che richiedono tempi lunghi che non sono compatibili con l'urgenza dei problemi attuali; o ancor meno affidare la questione del Mezzogiorno alla fatalità delle case da gioco, come si è discusso troppo abbondantemente questa mattina. mattina. Politiche attive per il Mezzogiorno per noi significa creare le condizioni perché le banche siano indotte ad operare di più e meglio nel Sud, a gestire meglio i fondi agevolati per il Meridione. Voi al contrario avete tolto al Mezzogiorno ogni strumento attivo a livello nazionale per sostenere gli investimenti delle imprese e siamo ancora in attesa, ad oggi, di conoscere dell'approvazione da parte del Governo delle risorse vere da destinare ai piani regionali per la spesa per il Sud. Voi vi siete chiesti: è meglio nascondersi sotto l'alibi del debito pubblico o far finta di risanare i conti pubblici con tagli alla cieca, che colpiranno i settori del Paese su cui al contrario si dovrebbe investire? La spesa pubblica è malata di inefficienza: solo nel 2008 le risorse inutilizzate ammontano a 13 miliardi e a 20 miliardi la parte della spesa che sfugge a ogni controllo. Noi diciamo che il contenimento della spesa pubblica non può prescindere da un'attenta e a volte anche impopolare opera di razionalizzazione, in cui è importante ridefinire le priorità nella distribuzione dei fondi pubblici e modificare l'ordine delle voci, eliminando quei comportamenti che la Corte dei conti nella sua ultima relazione annuale ha definito patologie da devianza. Infine, cari colleghi della maggioranza, voi vi siete chiesti: è meglio stare fermi o fare qualcosa? maggioranza, che non vi manca soltanto un progetto condiviso per il futuro del Paese, non vi manca soltanto una uniformità di proposte; vi manca qualcosa di più importante: il senso di responsabilità e il coraggio. Dietro l'ansia di correre dietro ai vostri sondaggi di gradimento e la ricerca di trucchi contabili per far tornare i conti, avete rinunciato ad analizzare ma soprattutto a capire la realtà in cui vive il nostro Paese. Alla fine avete iniziato a pensare anche voi che tutto sommato, con il pretesto di qualche *escort* in più o di processi brevi, è meglio tornare alle elezioni anticipate.

completiamo oggi il primo passaggio del disegno di legge finanziaria che sicuramente è una finanziaria anomala, di transizione verso la nuova legge di contabilità, che quindi rivedrà proprio la procedura con cui la si compone; una finanziaria che sappiamo essere ridotta negli importi perché la finanziaria vera è già stata fatta lo scorso anno e i saldi sono chiusi, tant'è che il maxiemendamento su cui ci siamo dilungati oggi tutta la giornata e anche nella giornata di ieri alla fine è

Una riforma vera sicuramente è quella del bicameralismo perfetto, che di perfetto a nostro avviso non ha un bel niente, tant'è che la discussione approfondita su temi importanti (pensiamo all'IRAP, alla cedolare sugli affitti e quindi anche alla detrazione per gli inquilini) adesso ci lascia un po' a bocca asciutta perché l'argomento sarà discusso alla Camera dei deputati

conseguente detrazione per gli inquilini, con un emendamento. Un'operazione del valore di svariate centinaia di milioni di euro va approfondita ed è il Governo che, alla fine, deve trovare la sintesi. Noi speriamo che si trovi questa sintesi entro la fine dell'*iter*

anzi di pagare per lavorare. Questa è la situazione in cui si trova un imprenditore che è in perdita: ha lavorato, non ha guadagnato e in più deve pagare le tasse. È evidente che questa è una stortura, per

anche perché non possiamo più sostenere in eterno questa divaricazione tra la spesa pubblica, che rimane costante, e le entrate, che invece sono legate al solo settore privato e quest'anno hanno avuto un calo molto rilevante.

l'impresa continua ad andare male e il calo del fatturato non è compensato da riduzioni di spesa, c'è la cassa integrazione, poi la mobilità ed infine i licenziamenti.

contrasto è stridente. Nella pubblica amministrazione non c'è la cassa integrazione, figuriamoci la mobilità e i licenziamenti. Prima o poi, questi due mondi ‑ quello virtuale della pubblica amministrazione e quello reale che invece la finanzia ‑ dovranno trovare necessariamente un accordo e un equilibrio. Come è possibile ottenerlo? Sappiamo tutti che è

veramente e approfonditamente è fare quelle benedette riforme che la Lega Nord propugna da anni e anni: non solo il federalismo fiscale, per la responsabilizzazione degli enti locali a tutti i livelli, ma anche

speditamente all'approvazione del riordino degli enti locali abolendo tutto ciò che si può abolire, semplificando tutto ciò che si può semplificare è assolutamente necessario, perché per forza di cose dobbiamo ritrovare un equilibrio fra la parte pubblica e la parte privata del Paese, che è quella che tutti i giorni rischia, quella che tutti i giorni non sa se tira su la "cler" e avrà nel cassetto i soldi a sufficienza per pagare i propri dipendenti, i propri operai, i propri impiegati. Questi due mondi devono necessariamente trovare un equilibrio e per noi l'equilibrio lo si può trovare semplicemente facendo queste drastiche e profonde riforme. potremmo mettere a posto la finanza pubblica e anche dare fiato alle nostre imprese private che fanno fatica a competere sui mercati internazionali, anche perché sappiamo tutti che con un calo della domanda che si registrerà stabilmente nei prossimi anni abbiamo bisogno di rendere più competitive le nostre aziende.

Dopo vengono le tasse. Le due cose, secondo noi, possono andare tranquillamente di pari passo: ridurre la burocrazia, sia come dimensione sia come inefficienza, e ridurre le tasse. Per farlo bisogna semplicemente fare le riforme: federalismo fiscale e riordino degli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, abbiamo osservato con curiosità e anche con attenzione in questi giorni di lavoro parlamentare il frenetico immobilismo con il quale maggioranza e opposizione si sono accinte all'opera di approvazione di questo disegno di legge finanziaria. Adopero un ossimoro, è ovvio, e forse potrei adoperare un'immagine: è stato come assistere a certe comiche della prima cinematografia, bianco e nero, senza sonoro. Non so se riesco a focalizzare il vostro ricordo. C'è una moltitudine di bombette, di grembiulini, di gente che si alza, scende, si siede, sale le scale, le ridiscende precipitosamente, si sposta da destra a sinistra e, ad un certo punto, il fermo immagine: è rimasto tutto identico a come era prima. Lì normalmente la sala scoppiava in una risata. Qui, in realtà, non c'è niente da ridere. questa finanziaria è assai più facilmente descrivibile; in realtà, descrive molto bene in quanto corrisponde al nulla, perché anche il nulla significa e descrive. E la prima valutazione che mi viene da fare è che certamente descrive una grave difficoltà e un serio infragilimento del Governo. Certo, se dovessi guardare ai numeri di molteplici votazioni, al di là del fatto che il Regolamento del Senato - e solo il Regolamento del Senato - equipara le astensioni ai voti contrari, dovrei dire che questo Governo è stato più volte politicamente battuto in quest'Aula. Perché questo poi è il punto. Ma io vorrei riferirmi a questa fragilità politica che si è manifestata certo in maniera molto vistosa con il sistema degli emendamenti che sono stati presentati da autorevolissimi rappresentanti di questa maggioranza. Erano emendamenti che probabilmente avevano dei difetti, mancavano talvolta di copertura oppure presentavano uno strumento che poteva considerarsi contestabile, ma erano una proposta di governo, erano una proposta di politica economica. E non è un caso che su una grande quantità degli oggetti e degli obiettivi indicati in quel sistema c'era una piena coincidenza con le proposte che venivano dall'opposizione. Questa, peraltro, che è possibile trovare, rispetto ai bisogni del Paese e rispetto, direi quasi, alle ovvietà delle necessità e dei bisogni del Paese, una coerenza tra le scelte e le posizioni della maggioranza e (*Segue* FINOCCHIARO*)*. La cedolare secca sugli affitti, il credito d'imposta, gli investimenti sulla ricerca, il taglio dell'IRAP, il fisco per le famiglie, gli investimenti sul lavoro, il Mezzogiorno: appunto, una proposta di politica economica per il Paese. Ma il nulla descrive, il nulla, ovvero nessuna proposta di politica economica descrive. E descrive un'altra cosa; questo è un altro degli elementi di fragilità, mi pare a questo punto, del Governo e della sua relazione con la sua maggioranza: descrive anche lo scolorimento di una identità politica della coalizione che governa il Paese, ma più propriamente della proposta politica del Presidente del Consiglio, che aveva certo caratteri identitari fortissimi, che si sono imposti in periodo elettorale e che lo hanno condotto a vincere le elezioni, caratteri identitari riconoscibilissimi, anche perché poi supportati da una capacità di propaganda e di proposizione pubblica molto efficace. Uno di questi tratti identitari assolutamente inequivocabili era quello della sicurezza dei cittadini, su cui la maggioranza ha basato la campagna elettorale e che è stato uno dei dei motori del successo della coalizione, vero o falso che fosse. Era falso, perché con questa finanziaria si completa un'opera che è cominciata nel 2008, dal primo giorno in cui avete iniziato a governare: sono stati tagliati 900 milioni di euro solo

sul magheggio, sull'illusionismo dei 100 milioni che mettete a disposizione, ma se anche fossero veri, è talmente ampia la sproporzione tra ciò che è stato tagliato e ciò che si mette a disposizione che, per una volta, vi direi visto che vedo continuamente, in tutte le occasioni esponenti della maggioranza e del Governo vantarsi dei successi nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata (sulla legislazione varata in questa legislatura noi rivendichiamo di aver dato il nostro apporto e contributo decisivo) forse è il caso di smettere di vestire così frequentemente e così palesemente le penne del pavone. Magari questi risultati sono dovuti al lavoro di quelle forze dell'ordine a cui non pagate gli straordinari e di quei magistrati che ogni giorno insultate Gruppo PD e del senatore Pardi).* Questo tanto per mettere un po' di ordine nelle questioni. E magari gran parte dei successi che il Presidente del Consiglio riscuote nelle zone terremotate sono dovute a quei vigili del fuoco a cui ancora lo straordinario per il terremoto d'Abruzzo non l'avete pagato. Tanto per ricordare qualcosa. Sicurezza: questo è il punto. Nel frattempo offrite alla discussione pubblica il disegno di legge Gasparri-Quagliariello. In proposito dico solo una cosa: mi augurerei che il Governo avesse il buonsenso di accogliere immediatamente la proposta che voglio fare in questa sede a nome del mio Gruppo, e cioè che, prima di aprire il fascicolo in Commissione, il ministro Alfano venga in Parlamento a farci una valutazione del numero di procedimenti che andranno al macero con questo provvedimento. *(Applausi dal merito, costituzionalità. Solo questo: quante centinaia di migliaia di processi penali andranno al macero. E poi, ovviamente, il capitolo forse più brillante con il quale dall'inizio della sua discesa in campo, nel 1994, il presidente Berlusconi ha voluto connotare la sua presenza politica sulla scena italiana: il taglio delle tasse. Non ce n'è traccia, vorrei essere molto chiara su questo. Sarebbe troppo semplice dire che il presidente Berlusconi aveva annunciato che avrebbe cancellato l'IRAP e qui sono stati respinti tutti gli emendamenti che erano stati presentati a riduzione dell'IRAP, e in particolare quelli del mio ha illustrato il senatore Morando, servivano tra l'altro a sostenere l'occupazione. Anche sulla vicenda dell'IRE, però, dovreste dire agli italiani - tanto se ne accorgeranno da soli - che gli state levando una frazione dell'acconto, ma gliela chiederete a saldo: li pagheranno tutti, Non sono sconti e saldi sulle tasse che questo Governo sta regalando agli italiani. Poi c'è il capitolo del prestigio dell'Italia e delle politiche internazionali. Allora spiegateci perché avete tagliato il fondo di finanziamento delle missioni internazionali, affidando alla ricerca spasmodica del Ministro dell'economia e delle finanze un capitolo così importante della politica internazionale e delle relazioni internazionali del nostro Paese. E diteci dove sono i soldi della cooperazione. Non c'è niente sulla famiglia, che pure è stato un altro cavallo di battaglia. Non c'è niente sulle imprese, che infatti se ne sono accorte e sono un po' nervose. Non c'è niente sulle Forze armate. In compenso avete privatizzato anche armamenti ed immobili, un grande *business*. Di questo torneremo a parlare nei prossimi giorni, perché è un capitolo troppo delicato per essere liquidato così brevemente. Quindi, scolorisce la stessa natura identitaria, la stessa fisionomia politica della coalizione di Governo. E, secondo voi, vi basta ancora, e per quanto tempo, solo l'immagine sia pure radiosa del Presidente del Consiglio? E poi, non fate finta di non capire: il *boom* economico descritto dal *premier* qualche giorno fa si scontra troppo duramente con i dati. Ho pregato i colleghi di segnalarmi quali imprese siano a rischio nel loro territorio: credevo di aver chiesto una cosa ovvia ed ovviamente i risultati sono stati difficili, difficili anche soltanto da leggere. Leggerò solo qualche dato, tanto per dare un'idea dell'intero Paese, della crisi che riguarda il sistema economico-produttivo dell'intero Paese. Comincio dalla Sicilia, dalla mia terra. La FIAT di Termini Imerese chiude. Nei cantieri navali sono tutti in cassa integrazione. Parliamo dell'Umbria? Il gruppo Merloni conta 2.800 posti a rischio. Parliamo di Bologna? Abbiamo 24.000 dipendenti con ammortizzatori sociali, 1.000 aziende a rischio di chiusura fino al 2010 e 570 a rischio chiusura a fine anno. Parliamo della Basilicata? I dati sono analoghi. Potrei continuare, potrei andare avanti. Non c'è più distinzione tra Regioni ricche e Regioni disagiate, come si diceva una volta. La crisi è crisi e sta provocando disoccupazione, espulsione dal mondo del lavoro, cassa integrazione guadagni cassa integrazione in deroga che stanno finendo e rispetto alle quali le Regioni che hanno fatto l'anticipazione non hanno visto ancora un soldo. Sono destini umani, sono famiglie, sono imprese. Voi dite sempre che non c'è conflitto sociale, perché questo è un Paese di gente seria. di gente seria. Credo che dovremmo anche ringraziare gli imprenditori italiani, e in particolare i piccoli e medi imprenditori che stanno tenendo una relazione vera con i propri lavoratori, perché loro sanno che da questa relazione e da quella permanenza dipende anche la sorte di quelle imprese e il benessere di un intero territorio. Non voglio essere pessimista, e neanche distruttiva. Il fatto che sia stato dichiarato inammissibile, come era giusto che fosse, l'emendamento sulla Banca del Sud non significa che noi non siamo pronti a collaborare ad una discussione vera sul credito nel Mezzogiorno, che è una delle questioni che dobbiamo certamente affrontare, e affrontare rapidamente. Ma una cosa vi voglio dire: non fate più finta di niente! Non è più possibile fare finta di niente. Siete un Governo legittimo, governate questo Paese in base ad un voto popolare. Noi vi chiediamo di avere la forza e l'umiltà di riconoscere qual è lo stato del Paese Paese ed anche la forza e l'umiltà di capire che, andando avanti così, la corda può spezzarsi e che non ci sarà vincolo dato dalla legge elettorale, dalla forza della *leadership* che potrà tenerla insieme, perché troppe sono le spinte, i bisogni, le necessità, talvolta addirittura l'urlo che viene dai territori e che comunque coinvolge tanti parlamentari di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che sanno che comunque dovranno rendere conto al popolo italiano di ciò che riusciranno a fare in questa fase della sua difficile storia.

*(PdL)*. Signor Presidente, se volessi fare la dichiarazione di voto sulla legge finanziaria per conto del Popolo della libertà con gli stessi toni polemici che ho sentito fino a questo momento, la cosa sarebbe oltremodo facile,

tutto l'impianto logico che ho ascoltato nelle dichiarazioni di voto è il seguente: signori del Governo, avete tagliato questo, questo e quest'altro, ma non avete tagliato le tasse e non avete aumentato adeguatamente un certo tipo di spese. È ovvio che sarebbe facilissimo governare diminuendo continuamente le entrate e aumentando le spese, ma ciò ovviamente non è possibile. allora questa fase finale delle dichiarazioni di voto per concentrarmi invece, com'è giusto da parte della maggioranza, su ciò che il Governo concretamente fa con questa finanziaria e su ciò che concretamente propone di fare nel prosieguo della stessa. tale ragione, senza dover per niente cedere alla demagogia, voglio cominciare a dire che questo è il primo passaggio della legge finanziaria e che ormai da due anni la stessa si inquadra in un complesso di provvedimenti economici e finanziari del Governo.

all'economia italiana, ha di recente promosso lo scudo fiscale, le cui entrate - è noto - saranno devolute interamente a spese per il sostegno e lo sviluppo dell'economia, oltre che a spese per le fasce più deboli della società, possano sentire meno i morsi della crisi. Non soltanto; voglio sottolineare che questo provvedimento si inscrive anche in altri importantissimi provvedimenti che il Governo ha assunto. Voglio solo ricordare a tutti i colleghi che sono intervenuti l'enorme disponibilità

che vengono da una situazione molto grave, non si aggravano più degli altri; in secondo luogo cresciamo nella media o meglio degli altri. Due aspetti cardine che dobbiamo stare attenti Pertanto il Governo continua a usare una politica di rigore nei conti pubblici e, allo stesso tempo, a cogliere tutte le opportunità per attendere il momento della ripresa; questo è il senso della politica del Governo. Voglio ricordare a tutti che anche in Germania, in Francia, vieppiù in vieppiù in Inghilterra e tanto più in Spagna la questione dei conti pubblici è ancora oggi la più importante tra quelle che i Governi devono affrontare, ed in questo quadro si inscrive questa legge finanziaria.

furono appostati circa 18 miliardi di euro per favorire i pagamenti della pubblica amministrazione in favore delle imprese. Certo, i crediti delle imprese sono di gran lunga superiori, ma intanto il Governo e questa maggioranza con i 18 miliardi in oggetto hanno contribuito alla circolazione della liquidità per per le imprese, uno dei momenti fondamentali per superare questa crisi. Ci sono poi alcuni provvedimenti che voglio ricordare. Innanzi tutto, questa finanziaria continua una norma importante, quella delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, edilizie, che è stata varata, va detto, anche con il concorso delle opposizioni quando è stata fatta e che si è rivelata una norma importante che continuiamo a finanziare proprio con questa manovra.

tale comparto abbiamo avuto il grande rifinanziamento del Fondo di solidarietà e la proroga delle agevolazioni contributive per gli agricoltori, che tutto il mondo meridionale e settentrionale richiede e che unifica il comparto dell'agricoltura. Vale lo stesso per la giustizia e la pubblica sicurezza. Abbiamo spiegato più volte che ciò che hanno detto i colleghi dell'opposizione non corrisponde a verità. Le risorse che vengono date alla sicurezza con questo emendamento sono

degli immobili confiscati alle organizzazioni mafiose per darli alla giustizia e alla pubblica sicurezza è un altro segnale vero di attenzione per la giustizia e per la pubblica sicurezza. *(Applausi

con coperture certe e strutturali, perché solo tali coperture possono dare i vantaggi che i cittadini richiedono con la diminuzione delle imposte. Alludo al dibattito sull'IRAP, a quello sulla cedolare secca, ma potrei citare anche il cuneo contributivo od altro.

la sfida che la maggioranza lancia all'opposizione è quella di evitare facili polemiche e di impegnarsi, come a tratti ha già fatto, su un percorso serio di risanamento dei conti pubblici e di sviluppo dell'Italia. Questo è il punto fondamentale di fronte al quale ci troviamo.

è la continuità della politica finanziaria ed economica di questo Governo che, per il momento, fa dell'Italia uno dei Paesi che meno ha usato fondi pubblici a causa della crisi. Non c'è paragone tra la tenuta dei conti in Italia e quella degli altri Paesi. L'Italia si pone il problema dello sviluppo e, nel contempo, quello della solidarietà sociale: ho citato la cassa integrazione ma potrei anche rifermi ad altro: ripeto che si sta concretamente evitando che i morsi della crisi ricadano sulle spalle di chi lavora. Mi pare un disegno organico, criticabile, migliorabile ma che certamente non può essere misconosciuto. Con questa serenità noi annunciamo il nostro voto favorevole alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Noi diciamo, e non lo nascondiamo, abbiamo fatto anche riforme di sistema come il federalismo fiscale, con il concorso determinante dei colleghi dell'opposizione, e la riforma del bilancio, che sarà definitivamente approvata presso questo ramo del Parlamento, sempre con il determinante contributo dell'opposizione. Anche queste grandi riforme contribuiranno al risanamento dei conti pubblici e allo sviluppo dell'Italia. Questo mi pare mostri la serietà della nostra impostazione. Questo è il livello del dibattito se fin d'ora non si accedesse ad inutili polemiche strumentali e ad uso giornalistico ma invece ci si impegnasse ancora, concretamente, sul terreno della politica, delle istituzioni e dell'economia, credo che renderemmo un servizio al Paese. E questo il Governo Berlusconi sta facendo in questo momento.

mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1791, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti formali che si rendessero necessari. Dichiaro aperta la votazione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per 1'anno finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge finanziaria 2010 approvato dal Senato della Repubblica, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente apportate nel corso dell'esame parlamentare. È da evidenziare che i suddetti effetti vengono considerati con riferimento alla ormai consolidata struttura del bilancio per missioni e programmi e, quindi, alle unità previsionali di base approvate dal Senato. In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per l'anno 2010 in termini di competenza e di cassa; al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010-2012 in termini di competenza, nonché al bilancio programmatico; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) ed agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri (Tabelle nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici.